Comunico che, in data 8 febbraio 2007, è stato presentato il seguente disegno di legge: *dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai Ministri per le politiche giovanili e le attività sportive, dell'interno e della giustizia:* «Conversione in legge del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, recante misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche» (1314). **Per comunicazioni

che è stato accusato di razzismo, revisionismo e revanscismo, siano francamente inaccettabili, soprattutto perché espresse dal massimo rappresentante istituzionale di un Paese amico. Un Paese che l'Italia ha aiutato nel percorso di integrazione europea; un Paese che da noi ha avuto tutto il sostegno possibile, anche nei momenti più difficili. Ritengo siano ancora più inaccettabili nel momento in cui si riferiscono a parole che il Presidente della Repubblica italiana ha espresso in una giornata importante, il «Giorno del ricordo», il «Giorno del ricordo», in cui il nostro Paese intende tributare un doveroso omaggio a tanti innocenti, vittime di una stagione di odi e di vendette. Credo che per queste ragioni sia necessario che anche il Senato della Repubblica possa discutere di queste dichiarazioni. Pertanto, sono a chiederle d'intervenire nei confronti del Governo e del Ministro degli affari

chiarire con precisione quali sono le verità storiche, per convincere gli amici croati che l'atteggiamento che il loro Presidente sta tenendo è profondamente sbagliato e per fare in modo che su questa vicenda ci sia anche una presa di posizione da parte dell'Istituzione che siamo qui a rappresentare.

In apertura di questa seduta, la prima all'indomani del 10 febbraio, giorno dedicato al ricordo dei martiri delle foibe, dell'esodo dalla propria terra di istriani, dalmati e fiumani, ritengo giusto e doveroso farmi interprete del sentimento dell'Assemblea del Senato, esprimendo il commosso ricordo per le tante vittime innocenti di allora e la vicinanza ai familiari di quanti furono così barbaramente assassinati e di coloro costretti a lasciare le proprie case, i propri paesi e le proprie città. Nei giorni scorsi abbiamo tutti ascoltato e condiviso le limpide e misurate parole del Presidente della Repubblica a cui, sicuro di rappresentare l'animo di tutta l'Assemblea, rinnovo un ringraziamento forte e sincero. L'istituzione del «Giorno del ricordo», grazie ad una legge approvata nel 2004 dal Parlamento, offre l'opportunità al Paese di fare memoria di una pagina terribile che ne ha segnato la storia nel secolo scorso. Una tragedia troppo a lungo dimenticata ed è bene riconoscere che sono stati commessi un grave errore e una ingiustizia verso quelle italiane e quegli italiani vittime di un odio ideologico ed etnico costato migliaia di morti e l'esodo per centinaia di migliaia di essi. Rinnovare il ricordo di quei drammatici eventi ci deve anche fortificare nella convinzione che non ci può essere un futuro comune tra i popoli se non all'insegna del riconoscimento reciproco, dell'amicizia, del superamento di qualsiasi barriera politica, culturale ed etnica e nella piena affermazione della libertà e della democrazia. Vi invito ad osservare un momento di raccoglimento.

sono gravi e che è giusto il richiamo che altri colleghi hanno fatto in quest'Aula.

Ricordo che a Roma, alcuni anni fa, è stata dedicata una piazza importante ai martiri delle foibe istriani e dalmati. Le affermazioni dell'altro giorno del Presidente della Repubblica, quando ha consegnato gli attestati e ricevuto i familiari degli italiani che dovettero abbandonare, in 350.000, quelle terre, riscattano finalmente il silenzio di cinquanta anni su italiani che hanno pagato con la loro vita la prima pulizia etnica in quei territori. Presidente, le sue sono parole che rappresentano e vogliono rappresentare l'intero Senato, ma noi siamo qui a voler ricordare ancora una volta con commozione quegli italiani che sono rientrati in Patria, che sono andati all'estero, che hanno onorato l'Italia avendola sempre nel cuore; tanti sono quegli italiani,

alla nostra interrogazione, che non rispecchia altro che le dichiarazioni del Presidente della Repubblica, che Alleanza Nazionale ha completamente condiviso. Presidente, credo sia mio dovere intervenire perché l'espressione che fa riferimento ad un lungo silenzio può essere equivoca. Vorrei spiegare ho vissuto quel periodo e quindi lo conosco direttamente - perché abbiamo coscientemente evitato di fare di quell'argomento un motivo che dividesse. Certamente, eravamo ispirati da due fattori. Innanzitutto, non doveva essere un motivo di polemica interna, perché i comunisti italiani non c'entravano niente;

più di un motivo di grandissimo contrasto, un clima di comprensione che guardasse al futuro e non al passato. Ritengo quindi che il silenzio sia stato più che giusto e che siano state molto opportune le parole dette.

degli italiani di quelle zone riteneva di dover guardare al futuro e non creare dei solchi che aggravassero ulteriormente la situazione.

per sottolineare un aspetto del problema che è stato focalizzato quest'oggi dal sindaco di Trieste, ha invitato ufficialmente il Presidente della Repubblica a rendere visita al Monumento nazionale della foiba di Trieste, inaugurato

che risultano - e ce ne sono molti ancora oggi - in proprietà delle Repubbliche sovrane succedute alla Repubblica sovrana di Iugoslavia. Si tratta di beni nazionalizzati che, per una serie di situazioni giuridiche, che in altro momento e in altra sede sono state e verranno illustrate, possono essere restituiti alla luce dei princìpi del diritto internazionale

in maniera puntuale, in apertura dei nostri lavori. Ritengo che nelle parole del Capo dello Stato e nell'annuncio fatto all'Aula in maniera solenne dalla Presidenza del Senato siano espressi tutti i nostri sentimenti e tutte le nostre volontà. Anche le integrazioni del presidente Andreotti servono a capire meglio quel fenomeno e a porlo nella luce che il Capo dello Stato ha già compiutamente

ora lettura del calendario dei lavori del Senato, come stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo di questa mattina. La Conferenza dei Capigruppo, riunitasi questa mattina, ha approvato all'unanimità modifiche ed integrazioni al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 22 febbraio. La seduta di domani mattina avrà inizio alle ore 10,30 - e proseguirà fino alle 13,30 - per consentire alle Commissioni affari costituzionali e bilancio tempi più ampi per la conclusione dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge recante proroga di termini legislativi. Nella giornata di domani, oltre al predetto decreto, sarà posto all'ordine del giorno l'esame di una relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari in materia di reati ministeriali. Pur tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 135-*bis* del Regolamento, il Presidente ha avuto mandato unanime dalla Conferenza dei Capigruppo di valutare, in relazione all'andamento dei lavori, quando procedere alla prima serie di votazioni con procedimento elettronico eccezionalmente anche nella seduta pomeridiana - al fine di favorire la più ampia partecipazione ai voti, in ragione del *quorum* della maggioranza assoluta richiesto per l'approvazione delle conclusioni della Giunta. In ogni caso, i senatori che non abbiano partecipato alle votazioni elettroniche potranno comunicare il proprio voto in modo palese ai senatori segretari fino alle ore 19, come prevede il richiamato articolo del Regolamento. Resta confermato, per giovedì mattina, l'avvio della discussione generale del decreto-legge recante recepimento di direttive comunitarie. Nel corso della stessa seduta avranno inoltre luogo comunicazioni del Governo sulle recenti operazioni antiterrorismo, cui seguirà un dibattito, senza voto di strumenti di indirizzo. I tempi saranno comunicati ai Gruppi. La prossima settimana, nella seduta antimeridiana di mercoledì 21 febbraio, il Ministro degli affari esteri renderà comunicazioni al Senato sulle linee di politica estera. I tempi della successiva discussione sono stati ripartiti tra i Gruppi, in modo tale da consentire la conclusione delle eventuali votazioni entro la fine della seduta antimeridiana, prevista per le ore 14-14,30. Nel corso della prossima settimana potrà inoltre proseguire l'esame dei due decreti-legge in calendario, per i quali si è proceduto alla ripartizione dei tempi tra i Gruppi.

o di chi ha solo saputo della sua eccezionale biografia, alla quale in questi giorni hanno reso omaggio le forze politiche e lo stesso Presidente della Repubblica, corre a quegli anni, all'inizio degli anni Settanta quando lei, donna già matura, fu testimone del suo tempo e illustre e coraggiosa protagonista della battaglia per i diritti civili degli ultimi, dei carcerati e, in prima linea, delle donne, per il divorzio e per ottenere la legalizzazione dell'aborto, dell'interruzione volontaria della gravidanza. Adele Faccio apparteneva ad un'illustre genealogia femminile. Nipote di Sibilla Aleramo, partigiana combattente nelle sue martoriate terre di confine contro il nazifascismo, studiosa e letterata. Io la conobbi - lo ricordo, anche se allora ero giovanissima - nel movimento femminista di Torino. Appartenevamo a pensieri e culture diverse, quando lei a Torino, insieme ad Adelaide Aglietta, fondò il Movimento di liberazione della donna. A Firenze fondò il CISA, mentre nelle grandi città italiane, specialmente quelle del Nord, si affermava la lotta per i consultori autogestiti. Da quella fase di battaglie, da quelle lotte aspre ed anti-istituzionali che lei nobilitò con la sua intransigenza, sino alla disobbedienza civile estrema e all'arresto,

riuscirono a portare a legalità, a legislazione, a produrre buone leggi sul divorzio, sull'aborto, difendendolo con il *referendum* del 1981. Questa stagione istituzionale, più solida, più di massa, che ha dato al Paese leggi buone ed equilibrate, porta però nella sua genesi, nel suo farsi, nel suo atto di nascita, anche il ricordo di quelle lotte solitarie estreme che Adele Faccio, insieme ai suoi compagni radicali e a molte donne, combatté. Ricordo agli ambientalisti che Adele fu anche fondatrice dei Verdi Arcobaleno e che nell'VIII legislatura si fece propugnatrice di molte leggi sui limiti dello sviluppo, sullo sviluppo sostenibile e sui nuovi problemi ambientali.

laddove si propone che non solo i suoi compagni radicali, ma tutti gli ambientalisti e tutto il mondo della politica si diano da fare in suo ricordo con qualcosa di concreto, che trasmetta la sua cultura e i suoi insegnamenti, soprattutto ai più giovani.

che ho avuto l'onore di conoscere in Parlamento e di apprezzare per le sue capacità di affrontare i problemi, anche più delicati e difficili, con uno spirito aperto, non fazioso, più desideroso di convincere che di imporre le proprie opinioni, come dovrebbe sempre essere. Adele Faccio era una donna straordinaria per il modo in cui era capace di affrontare, in tempi difficili e diversi (mi permetto di dire anche peggiori di quelli di oggi, per quanto attiene alla condizione femminile), i valori di una società che ha bisogno di una grande e nuova forza, che stabilisca l'equilibrio nei rapporti civili, sociali ed umani nel nostro Paese. Era una donna coraggiosa, non temeva l'impopolarità; quello che doveva dire lo diceva sempre, con chiarezza e con il senso delle proprie convinzioni, nel rispetto di quelle altrui. Credo sia una parlamentare che va ricordata come esempio di come ci si deve comportare in Parlamento: con rispetto e con forza. Forza delle proprie convinzioni, rispetto di quelle degli altri. Ecco come io ricordo Adele Faccio. anch'io per unirmi al ricordo di Adele Faccio. L'ho conosciuta abbastanza bene: era una donna dolcissima nei rapporti amicali, di grande discrezione e di grande affettuosità; rigorosissima nei rapporti politici e di principio. Rigorosissima prima di tutto con se stessa; un'etica assolutamente di grande rigore e di grande precisione. Di lei posso dire di aver apprezzato tutte le lotte che ha iniziato e che ha fatto, mettendo sempre in gioco se stessa e tutta la propria vita. Quello che posso dire è che in questa temperie ciò che apprezzo di più è stata la sua capacità di sopportare anche dolorose vicende familiari (il figlio) e la sua capacità di sottrarsi all'impero mediatico. Le persone che sono capaci di vivere con discrezione un periodo di oscurità sono oggi, a mio parere, dei modelli assolutamente inarrivabili e rari. Adele Faccio è stata anche questo.

l'onorevole Luigi Memmi, che da parlamentare della Repubblica e da profondo conoscitore dei problemi del Mezzogiorno d'Italia si applicò non poco, nel Parlamento nazionale prima e, per un lungo periodo, come sindaco della sua città, Casarano, che fu catalogata, grazie anche alla sua azione, tra i primi cento Comuni della Repubblica italiana, quelli che più degli altri avevano conseguito progresso e sviluppo per le genti del Mezzogiorno nei primi cinquant'anni della Repubblica. Al suo impegno nella Commissione bilancio e per la legislazione in materia di bilancio va il nostro grato ricordo e affettuoso pensiero.

a portare all'attenzione dei colleghi che il provvedimento che andiamo a discutere oggi non solo ha un significato importante sotto il profilo economico-culturale, ma anche un forte rilievo politico. Il rilievo economico-culturale è dato dalle prospettive di apertura del mercato cinese alla produzione cinematografica italiana, nonché dalle potenzialità che tale *partnership* è in grado di offrire alla produzione italiana. Infatti, si deve tener conto, da un lato, della vivacità della produzione cinematografica cinese, che, come i colleghi sanno, nel recente passato ha conseguito significativi e importanti successi e riconoscimenti nelle manifestazioni culturali internazionali e anche in quelle più significative del mondo occidentale

Sotto il profilo politico, lo ritengo importante perché bisogna tener conto che la ricca produzione ufficiale è accompagnata da una significativa produzione cinematografica non ufficiale da parte di operatori cinesi che, però, purtroppo, non possono diffondere le loro opere *in loco* perché soggetti a pesanti restrizioni. Questo accordo, dunque, rende auspicabile e probabile che da un'intensificazione della cooperazione culturale in questo campo con l'Italia ci sia, come risultato ineluttabile, una maggiore apertura di quel Paese in termini di rispetto dei diritti civili e politici; quindi, dalla coproduzione cinematografica deriverebbe una contaminazione positiva sul piano dei diritti. Il provvedimento, nello specifico, propone di realizzare un importante quadro normativo per lo sviluppo delle relazioni culturali tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare cinese, tramite la facilitazione della produzione in comune di film che, per le loro qualità artistiche e tecniche, possono contribuire alla maggiore conoscenza reciproca ed essere competitive dal punto di vista commerciale sia nei rispettivi territori nazionali che in quelli dei mercati terzi. Nel merito, l'accordo precisa il significato tecnico dei film in coproduzione e stabilisce che ogni film coprodotto goda degli stessi vantaggi dei film nazionali. Vengono poi individuati i requisiti che i produttori devono possedere, fissando al 20 per cento del totale del costo del film l'apporto minimo al progetto di coproduzione, e si stabilisce che il personale artistico e tecnico impiegato nella coproduzione debba essere di cittadinanza italiana, inclusi ovviamente i Paesi membri dell'Unione Europea, o cinese, inclusi i cittadini di Hong Kong o delle Regioni ad amministrazione speciale come Macao, e che tale personale è tenuto a rispettare la legislazione vigente, gli usi, i costumi e il credo religioso del Paese in cui le riprese hanno luogo. Ulteriori norme del provvedimento autorizzano poi l'ingresso di cittadini dell'altro Paese e la temporanea importazione di attrezzatura tecnica cinematografica nel territorio dell'altro Stato contraente, nonché lo svolgimento di riprese in Paesi terzi, laddove la sceneggiatura o l'azione del film lo renda necessario. Alla collaborazione e alla negoziazione tra i coproduttori sono quindi rimesse sia le decisioni riguardo all'accesso dei film in coproduzione ai festival internazionali, sia la ripartizione dei proventi derivanti dai diritti d'autore, che ovviamente appartengono a entrambe le parti contraenti. Rilevo, inoltre, per fornire informazioni ai colleghi, che l'Accordo dispone che i film coprodotti debbano essere esaminati ed approvati dalle autorità competenti dei due Paesi individuati dall'Accordo e precisa che gli stessi possano essere distribuiti e proiettati in pubblico all'interno e all'esterno di ciascun Paese solo dopo il rilascio del relativo permesso da parte delle relative autorità competenti, le quali, in base all'Accordo, con un successivo scambio di Note, provvederanno a fissare le norme di procedura per la coproduzione nel rispetto della legislazione vigente in ciascuno dei due Paesi.

anche a causa del numero elevato di abitanti. Di fronte a tale situazione, che credo sia assolutamente innegabile, vi sono due atteggiamenti possibili: quello della chiusura e quello del dialogo

con il voto da parte di un organismo che non è governativo, ma che indubbiamente è a suo modo rappresentativo di una vasta realtà, per l'assegnazione delle Olimpiadi del 2008 proprio alla città di Pechino. Pechino. Valutando i risultati che queste aperture dovrebbero avere generato, credo non si possa essere soddisfatti. La maggior parte delle organizzazioni che si occupano di diritti umani

siano state introdotte, almeno in teoria, norme di maggiore garanzia o, sarebbe più giusto precisare, di minore violazione dei diritti umani. Mi riferisco a quanto è stato proposto, per quanto riguarda la pena di morte, ad esempio per il diritto di appello a un tribunale, ad una corte diversa da quella che ha già decretato la condanna a morte di una persona;

Governo contro la droga o per l'accettazione di comunità con culture diverse dalla nostra), vengono fatte a suon di condanne a morte. Se la campagna è contro la corruzione, è necessario che ogni provincia od ogni distretto esibisca il suo adeguato numero di esecuzioni che vengono attuate con metodo brutale e sommario, a volte con processi che di fatto non sono neanche tali. Legaranzie, peraltro scarsissime, vengono invece attuate soltanto al di fuori di queste campagne. Pertanto, può accadere che per l'identica fattispecie di reato

non si sarebbe persa occasione, ad esempio nella relazione con cui il Governo presenta alla Camere il Trattato per la sua ratifica, per ricordare la necessità di superare quell'odioso regime che, infatti, fu superato in modo del tutto pacifico. Qui, invece, mi pare che in questo, come in molti altri casi, non si perda occasione piuttosto per

generare un'osmosi tra la nostra cultura, basata innanzitutto sulla libertà, e quella, in particolare cinematografica, cinese,

del mondo cinese che potrebbero dare luogo a film straordinari per le problematiche da presentare agli spettatori (che naturalmente ci si augura sempre siano molti) delle opere cinematografiche prodotte: si potrebbero, ad

uccise indirettamente attraverso la generazione di carestie artificiali, che in Italia venivano esaltate sotto l'etichetta del grande balzo in avanti di colui che si chiama sempre, con sussiegoso rispetto, il presidente Mao, uno dei più feroci dittatori che mai abbiano

da un giorno all'altro, con tre giorni di preavviso, per costruire meravigliosi impianti che impressioneranno i visitatori che, tra poco più di un anno, si recheranno in Cina per partecipare ed osservare questo grande avvenimento sportivo.

il 27 novembre 2006, il vicepresidente della Casa della cultura tibetana in Italia ha inoltrato, alla nostra ambasciata a Delhi, una formale richiesta di concessione dei visti per un periodo di 30 giorni ad una compagnia teatrale, un gruppo composto di 19 elementi di origine tibetana che hanno chiesto di venire nel nostro Paese perché invitati da una serie di enti, parecchi dei quali sono enti locali che hanno aderito che hanno aderito all'iniziativa "Amici del Tibet". In molti municipi ed in molte sedi provinciali è esposta la bandiera del Tibet,

di una coproduzione cinematografica. Purtroppo, a questi artisti è stato rifiutato, dalla nostra ambasciata a Delhi, la concessione del visto con delle giustificazioni un po' bizzarre: parrebbe che queste persone

ai novanta anni, forse con eccezioni che si potrebbero avere nel caso di qualche vegliardo che venisse comunque nel nostro Paese. Si tratta, inoltre, di una preoccupazione bizzarra, visto che non si ha notizia di tibetani, siano essi di nazionalità cinese o di nazionalità indiana, che abbiano violato le leggi sull'immigrazione. Aggiungo che è ulteriormente bizzarro che ci si preoccupi del rischio migratorio di un gruppo di 19 artisti quando in ogni altro aspetto dell'attività di questo Governo si fa di tutto invece per incoraggiare l'immigrazione, specialmente se clandestina. Mi riferisco a tutti i vari provvedimenti che costituiscono delle sanatorie di fatto o delle

del perché viene negato il visto a questi artisti tibetani che vorrebbero venire nel nostro Paese, invitati da istituzioni, che, tra l'altro, hanno anche stanziato del denaro, contando sull'ovvia concessione di tali visti. Non vorrei che il vero motivo che osta alla concessione dei visti sia il mantenimento di buoni rapporti con la Cina, che evidentemente preferisce negare la realtà dell'etnia, della cultura, della religione e diremmo anche della nazione tibetana e non gradisce che questo nome, questa cultura e questa religione vengano in alcun modo diffusi. A fronte di una risposta del Governo allora sentirmi meno a disagio nel votare tale provvedimento, altrimenti non riesco a capire perché incoraggiare il cinema e invece tenere fuori degli artisti che vengono invitati dagli enti locali. Altrimenti credo che non possiamo essere seri quando che nei contatti con la Cina e le autorità cinesi li si incalza, li si esorta e li si richiama al rispetto dei diritti umani. Il pragmatismo cinese, e non soltanto quello cinese per la verità, perché forse è un pragmatismo di molti regimi totalitari, è tale per cui possono benissimo ascoltare con pazienza il fervorino sui diritti umani e poi infischiarsene completamente e andare avanti. Ma allora o qui c'è un comportamento coerente, continuativo e serio oppure sarebbe meglio lasciar perdere i fervorini o o far finta di agire per il rispetto dei diritti umani. Qui non parliamo di cosucce: parliamo di 10.000 esecuzioni capitali l'anno, forse, perché neanche si può sapere la cifra. Parliamo di un popolo che si sta cercando di cancellare dal punto di vista della sua identità: c'è stata una cinesizzazione del Tibet, a fronte di 6 milioni e mezzo di tibetani ci sono sette milioni di cinesi che sono stati introdotti, di fatto quasi deportati in alcuni casi, per cinesizzare quella regione. Abbiamo una situazione di violazione sistematica dei diritti umani, con centinaia di migliaia di persone che si trovano nelle carceri per le loro convinzioni religiose, politiche o filosofiche; non possiamo far finta di nulla. Dunque, dobbiamo essere coerenti ed agire su tutto, a cominciare da questi piccoli accordi e scambi culturali.

colleghi, le relazioni culturali tra l'Italia e la Cina stanno acquisendo di anno in anno una consistenza sempre maggiore non solo dal punto di vista economico e politico, ma anche in termini di immagine internazionale del nostro Paese in Cina e viceversa. Lo spettacolo, ed in particolare il cinema,

ad aumentare, quanto meno a far crescere, la coscienza nei cinesi dei diritti umani. Quindi, ben venga questo accordo. Sempre più di frequente ci capita di vedere film provenienti dall'Oriente o girati nell'Est del mondo. Tra gli esempi più recenti abbiamo il film «La stella che non c'è» di Gianni Amelio, prodotto da RAI-Cinema, un ampio *cast* quasi esclusivamente composto da attori cinesi. La pellicola è stata tra le opere italiane in programma durante uno degli eventi di maggiore rilevanza internazionale degli ultimi mesi. Mi riferisco all'iniziativa italiana «Il cinema esplora l'Italia», organizzata da Cinecittà *holding* e promossa dal Ministero degli affari esteri e dalla Direzione generale per il cinema del Ministero per i beni e le si è svolta a Pechino e Shangai, dove per due settimane, dal 17 al 29 maggio, 30 lungometraggi del cinema italiano sono stati proiettati nelle sale cinematografiche più più prestigiose delle città cinesi, alla presenza di una delegazione di esponenti del mondo dello spettacolo (attori, produttori e distributori) tutti di alto livello. Un evento che per 15 giorni è riuscito a catalizzare l'attenzione del popolo cinese sul cinema e, attraverso di esso, sulla cultura italiana in ogni sua peculiarità regionale. Questi sono solo alcuni esempi della presenza italiana in Cina; un Paese la cui industria cinematografica ha dimostrato, nell'anno appena conclusosi, una capacità di sviluppo rapido ed intelligente, riuscendo ad imporsi nel mercato artistico globale. Nel 2006 i film di produzione nazionale sono aumentati di più di 300 unità rispetto all'anno precedente e le pellicole cinesi hanno ottenuto 44 premi nei *festival* internazionali, tra cui il prestigioso Leone d'Oro a Venezia. Alla crescita quantitativa si aggiunge quella qualitativa, che ha portato l'industria del cinema cinese al suo primo grande traguardo: uscire dai suoi confini ed arrivare in ogni parte del mondo. Cito, a titolo di esempio, il film «Hero» del pluripremiato regista Zhang Secondo le più recenti statistiche, l'intero territorio nazionale è arrivato a contare attualmente più di 1300 sale con oltre 300 schermi grazie ad una politica di diffusione cinematografica realizzata attraverso l'ampliamento della dimensione della copertura nelle proiezioni. Nel 2006, 16 zone sperimentali di otto province e regioni hanno proiettato 190 film con oltre 50 milioni di spettatori raggiungendo anche le zone rurali. L'Italia e la Cina rappresentano due Paesi che insieme possono realizzare di più, e sempre meglio, grazie anche a questo accordo bilaterale di coproduzione cinematografica che faciliterà lo spostamento delle persone coinvolte e del materiale necessario allo svolgimento delle riprese accordo incoraggerà, sosterrà e diffonderà le attività di coproduzione attraverso le rispettive autorità cinematografiche nazionali. È un accordo prezioso, che porterà enormi benefici non solo economici, ma anche culturali.

ci accingiamo a ratificare un accordo di coproduzione cinematografica. L'arte cinematografica è espressione di cultura e di libertà. Proprio in ragione della libertà di espressione, dobbiamo essere veramente preoccupati,

Per quanto riguarda la libertà di stampa è apparsa recentemente, anche su alcuni quotidiani italiani,

determinerebbe una parziale cancellazione di questi punti. Da tale parziale cancellazione potrebbe derivare una conseguente chiusura del giornale quando si dovesse arrivare all'azzeramento di questi punti. Questa è, a mio avviso, una forma di censura permanente, di controllo dell'espressione dei giornalisti che non può essere accettata dalle coscienze e dai concetti fondamentali di democrazia e libertà. È in ragione di questa situazione che l'organizzazione *Reporters sans frontières* afferma che nelle carceri della Repubblica popolare cinese

che sono imprigionati in ragione della loro posizione, cioè per via di quanto hanno espresso sui loro giornali.

quando, in occasione di un *question time,* avevo particolarmente evidenziato la questione della libertà religiosa nella Repubblica popolare cinese. Questo è un tema su cui chiedo al Governo di mettere in atto

alla capacità di determinare un percorso volto alla promozione e alla tutela dei diritti umani. Infatti, come ho detto

che ha permesso a questa Camera di istituire una Commissione speciale per la promozione e la tutela dei diritti umani, tali diritti non sono sono qualcosa che può essere oggetto di interferenza nella sovranità di uno Stato, ma sono dei principi, dei valori fondamentali che attengono il diritto inviolabile della persona umana.

ad un grosso sviluppo del sistema economico cinese, cui non è corrisposto un altrettanto rispettoso

un sistema nefasto a catena: peggio andrà in Cina, sempre peggio andrà sui nostri territori. l'impegno che chiediamo al Governo è proprio di far rispettare i diritti umani in Cina, che vuol dire avere maggior rispetto per i sistemi produttivi italiani ed europei che questi diritti, già da molto tempo, riconoscono.

il significato politico importante degli interventi di alcuni colleghi, nonchè degli ordini del giorno del senatore Pianetta e del senatore Divina.

Naturalmente, nell'intervento c'è stato un carico di giudizi storici epocali su cui poi si potrebbe aprire una discussione, fermo restando che

partecipare al voto di questo provvedimento, è che una *partnership* produttiva su temi culturali e su produzioni culturali ed intellettuali, anche di qualità, fa partire una contaminazione che, insieme a tante altre che cercheremo di cogliere - per cogliere anche le opportunità economiche che il mercato cinese offre in tanti settori - non possono che far bene

parere conforme a quello del relatore in merito agli ordini del giorno, sui quali però farò alcune proposte di riformulazione del dispositivo per renderli anche più efficaci e più coerenti. più efficaci e più coerenti. Il Governo è profondamente convinto che quest'accordo di coproduzione cinematografica tra la Repubblica popolare cinese e la Repubblica italiana intenda promuovere scambi e facilitare coproduzioni e quindi si muova all'interno di una stagione positiva di rapporti fra il nostro Paese e la Repubblica popolare cinese; recentemente, le due visite, quella del primo ministro Prodi a settembre dello scorso anno, seguita dalla visita del ministro degli affari esteri D'Alema, hanno permesso di costruire e consolidare una forte *partnership* strategica tra i nostri Paesi. In particolare, sono sostanzialmente quattro i settori sui quali abbiamo avuto la possibilità di siglare importanti intese, che aprono ad una grande cooperazione economica, commerciale, culturale, scientifica e politica fra il nostro Paese e la Repubblica popolare cinese:

Il nostro Governo è convinto che dobbiamo essere in grado (l'Italia, l'Europa, la comunità internazionale) di includere la Repubblica popolare cinese in contesti condivisi; questo è stato il caso dell'Organizzazione mondiale del commercio, ma voglio richiamare un altro fatto importantissimo: il dialogo strutturato tra Unione Europea e Repubblica popolare cinese sui diritti umani, che mi pare esattamente il contesto nel quale l'Unione Europea

porterà sempre più la Repubblica popolare cinese, come detto, in contesti di condivisione e quindi anche di condivisione di una cultura del diritto e della democrazia che noi auspichiamo, dobbiamo favorire e mettere anche in cantiere azioni concrete per favorirne le sviluppo e il processo.

da riformulare nel seguente modo: «Richiede al Governo di mettere in atto nelle sedi e nei modi opportuni azioni che possano contribuire a favorire nella Repubblica popolare cinese lo sviluppo delle fondamentali libertà di ogni persona, con particolare riferimento alle azioni già intraprese all'interno del dialogo strutturato Unione Europea-Repubblica popolare cinese sui diritti umani».

«Impegna il Governo ad attivarsi affinché ogni iniziativa di carattere economico e culturale nei confronti della Repubblica popolare cinese sia accompagnata da una verifica costante del rispetto dei diritti umani anche nel quadro delle azioni già intraprese all'interno del dialogo strutturato Unione Europea-Repubblica popolare cinese sui diritti umani». Questa proposta vuole dare coerenza rispetto ad un'azione molto strutturata e molto chiara che è già in atto.

chiedo scusa per la ripetizione, non avendo ricevuto la parvenza di una risposta - un gruppo concreto di 19 artisti tibetani che ha chiesto di venire in Italia. A questo gruppo è stato rifiutato

che quando si viene al punto c'è di fatto disattenzione; è inutile dire che si incalza, è inutile dire che si esorta se poi dal punto di vista pratico pratico la nostra ambasciata a Delhi, per questioni formali sicuramente ineccepibili, impedisce questo piccolo, vero scambio con una realtà realtà tibetana che non fa comodo al Governo della Repubblica popolare cinese, ma che esprime la cultura di un Paese, di una Nazione che è stata inglobata con le armi, con la violenza, con la pulizia etnica, con la repressione religiosa, ideologica, e persino demografica

Malan, il parere da lei citato sulle perplessità legate ai rischi di immigrazione clandestina che, al momento, hanno portato la nostra rappresentanza diplomatica a New Delhi, in India, a negare quella richiesta di visto.

non ritenessimo che sussistano quei rischi, non avremmo alcuna obiezione alla concessione di un visto, peraltro per un periodo di tempo limitato, ad una compagnia teatrale che svolge un'iniziativa di promozione culturale, tra l'altro patrocinata da alcuni importanti enti locali.

*Il Senato approva

così difficile e complessa a livello internazionale, il dialogo culturale, il dialogo sulle arti e con le arti, è fondamentale, è un punto essenziale. La coproduzione cinematografica con la Cina

i diritti umani siano punti essenziali per lo sviluppo della democrazia nel nostro Paese, penso sia opportuno votare a favore della ratifica dell'Accordo al nostro esame, perché mi sembra un passo in avanti nei rapporti con questo grande Paese con cui dobbiamo comunque fare i conti.

necessario invitare tutti coloro che parlano della Cina a tener conto delle condizioni tutte particolari Noi abbiamo un tono didattico e non teniamo conto delle notevoli trasformazioni in meglio che sono avvenute, qui è citato

dal Governo e approvato dalla Commissione affari esteri sentito il parere della Commissione bilancio. Si sottolinea come l'impegno del nostro Paese a sviluppare l'attività nel campo della ricerca, della scienza e della tecnologia figura tra gli obiettivi principali di questa nostra fase politica, economica, sociale, ben sapendo tutti quanto siano gravi ancora i ritardi del Paese che permangono al riguardo

In particolare, appare rilevante l'interesse dell'Italia ad espandere la cooperazione su questi temi con la Repubblica popolare cinese,

risulta uno strumento adatto a far compiere un ulteriore salto di qualità alla cooperazione bilaterale. Tra l'altro, signor Presidente, onorevoli colleghi, l'Accordo di cui si sta

Nel frattempo, dal 1998 in poi, in attuazione del primo Accordo siglato con la Repubblica popolare cinese, anch'esso di antica data, firmato il 6 ottobre 1978 dal quarto Governo Andreotti, ottobre 1978 dal quarto Governo Andreotti, la cooperazione bilaterale fra l'Italia e la Cina ha potuto giovarsi delle biennali riunioni della Commissione mista e della firma di Protocolli esecutivi di quell'Accordo, l'ultimo dei quali

stata approvata la mozione del senatore Andreotti per l'istituzione di una Commissione sui diritti umani. Ho riletto quanto è stato detto in quell'occasione: curiosamente, sono stati menzionati molti Paesi e molti casi concreti di violazione dei diritti umani, ma di Cina hanno parlato solo due senatori di Alleanza Nazionale e due senatori di Forza Italia. Questo non vuol dire che gli altri intervenuti non avessero presente la situazione; gli altri senatori hanno parlato del Brasile,

della feroce dittatura presente in Birmania e della gravissima situazione del Darfur, in Sudan. Credo che faremmo torto ad un minimo di conoscenza degli affari internazionali se non ricordassimo che la dittatura birmana è appoggiata dal Governo della Repubblica popolare cinese

discussione che si è svolta la settimana scorsa nell'approvare la Commissione sui diritti umani alle ratifiche di oggi non dovrebbe essere troppo brusco. Nella

risale al lontano 1998. Credo che non sia un caso se, dopo quasi nove anni, esso non è ancora stato ratificato. Ricordo che nella scorsa legislatura abbiamo smaltito tutto l'arretrato che avevamo trovato all'inizio della legislatura per quanto riguarda la ratifica di Accordi e Trattati internazionali e che abbiamo ratificato la grandissima maggioranza degli Accordi intervenuti nel corso del quinquennio.

il tempo passò e si giunse alla fine della legislatura nel 2001, senza arrivare alla ratifica, all'approvazione da parte di entrambe le Camere, anzi neppure da parte del Senato in Aula. scorsa legislatura si è fatto un passo in più, cioè l'approvazione al Senato, ma alla Camera si ritornò in Commissione quando già il provvedimento era in Aula, e dai resoconti sembra di capire per la stessa ragione. credo che dobbiamo porci veramente il problema di questo Accordo di cooperazione. Cito anche che, tra i campi di

dell'espianto di organi dai condannati a morte, sicuramente dopo l'esecuzione, ma non è escluso, da coloro che si occupano dei diritti umani, che a volte avvengano addirittura prima della morte. Abbiamo la testimonianza di un medico cinese, che ovviamente non vuole essere nominato, dell'aprile del 2006, il quale dice: «Una volta che il tribunale dà il suo consenso, i medici possono andare sul campo dove vengono svolte le esecuzioni, aspettano in un furgone sterile e raccolgono l'organo immediatamente dopo l'esecuzione. Tali esperienze causano un forte *shock* morale e mentale a molti chirurghi, perché i prigionieri di solito non muoiono immediatamente dopo essere Ma i chirurghi devono agire rapidamente perché gli organi abbiano i dovuti requisiti di freschezza» (usa proprio la parola «*freshness*»). In qualche modo «i medici sono parte dell'esecuzione», perché è chiaro che, una volta prelevati gli organi vitali, il condannato, benché non colpito a morte dallo dallo sparo che viene usato per giustiziarlo, evidentemente non può più vivere. Dice ancora: «Questo è troppo per molti giovani medici da accettare

dal punto di vista formale, cioè vengono presentati alcuni miglioramenti, ma di fatto si vada vada avanti verso una maggiore efficienza di questo sistema mostruoso che assomma il peggio del comunismo con il peggio del capitalismo, cioè la totale mancanza di rispetto per gli individui, per le comunità e per le etnie locali, per le religioni, per la libertà di opinione e anche uno sfruttamento scientifico, totale fino alle estreme conseguenze, come quella di predare gli organi ai condannati a morte, in punto di morte. A fronte di tutto ciò vengono presentati dei provvedimenti che sembrano venire un poco incontro agli appelli a favore dei diritti umani che vengono talora presentati, ritengo con scarsa convinzione e anche con scarsa fiducia (questo credo sia pienamente giustificato). Per esempio, per quanto riguarda la predazione degli organi, degli organi, è stata approvata una legge che stabilisce che ci voglia il consenso del cosiddetto donatore; questo però implica che il donatore sia vivo; quando il donatore è morto, evidentemente, il suo consenso non può più essere espresso e neppure negato. In questo caso, non una legge, ma una norma di rango inferiore stabilisce che sia la famiglia a poter disporre disporre dell'eventuale autorizzazione all'espianto degli organi. Credo, però, che il complesso della situazione politica e sociale, nella pratica, impedisca alle famiglie di esprimere un reale e sereno

di furto e di rapina, naturalmente per omicidio e così via; soprattutto, essa viene applicata con grande rapidità, senza garanzie processuali e ancora oggi senza possibilità di presentare appello ad un tribunale diverso da quello che ha pronunciato la sentenza di morte. Allora, di fronte ad una situazione di questo genere,

cercato di stabilire con la realtà produttiva, politica e sociale cinese (alla fine interamente controllata dal Partito comunista cinese), avesse ottenuto qualche risultato concreto. In realtà, abbiamo chiesto poco e ci si accontenterebbe di qualcosa di simbolico. fatto un appello, che io ho anche firmato, a favore dell'avvocato Gao Zhisheng, un attivista dei diritti umani che è stato imprigionato e che era ancora in prigione proprio quando il presidente Prodi, con la foltissima delegazione che lo accompagnava, si trovava in Cina.

presto), approfittando del grandissimo numero di cinesi ancora completamente tagliati fuori da qualsiasi tipo di benessere, sta accumulando un'enorme potenza finanziaria oltre che economica e produttiva che non esita ad usare in tutti i Paesi, in particolare in Africa, o anche per influenzare l'informazione e la politica occidentale. Allora credo che, di fronte a questa realtà, non possiamo far finta di niente. Ascolterò le repliche, ma francamente non mi sento in coscienza di dire sì a questo provvedimento. La fiducia data al Governo cinese nel 1998 e - torno a ripetere - nel 2001 quando sono state assegnate le Olimpiadi a Pechino, mi sembra che sia stata incamerata dando in cambio pressoché nulla: dei provvedimenti che di fatto non vengono applicati e che in gran parte addirittura non sono stati neppure approvati.

soltanto per ragioni politiche, di maggioranza o di minoranza. Stiamo parlando dei diritti umani in Cina e la cosa ha un'importanza immensa; è, questo, un argomento delicatissimo, che oltretutto sta a cuore proprio a quelli di noi che si sono sempre battuti per i diritti umani, da una parte e dall'altra, sotto qualunque denominazione politica.

firmai con il ministro degli affari esteri cinese, Chou En-lai, un accordo di collaborazione cinematografica. Succedono cose del genere: allora ero soltanto il direttore dei programmi culturali della RAI, però non c'era una rappresentanza diplomatica italiana e il Governo cinese, ansioso di avere delle relazioni, mi promosse, durante un viaggio di giornalisti italiani in Cina, al rango di interlocutore, visto che io chiedevo specificatamente, nell'incontro con Chou En-lai, la possibilità di girare documentari e film in Cina (in quel momento lo stavo chiedendo a nome della RAI). Ebbene, non solo è stato firmato quel protocollo nelle condizioni più strane, cioè tra un Ministro degli affari esteri e un non membro di Governo, ma è stato dato seguito a quell'accordo e ne è seguito - vi ricorderete - il film di Michelangelo Antonioni Non sto parlando del provvedimento appena approvato, cioè dell'accordo di coproduzione cinematografica, sto parlando dei rapporti con la Cina, e potete immaginare quanto i diritti umani fossero rispettati in quel momento. Ebbene, Michelangelo Antonioni ha potuto girare il suo film in Cina, perché in quel momento è coinciso con un interesse che la Repubblica popolare cinese, e in particolare la parte rappresentata da Chou En-lai, aveva, e il film è stato Ricorderete anche che il film è stato drammaticamente sconfessato e condannato dalle autorità della Repubblica popolare cinese e da quella che poi sarebbe stata definita la «Banda dei Quattro». Però è stato fatto e ha girato il mondo, gli Stati Uniti d'America; credo che 186 televisioni nel mondo lo abbiano trasmesso. Ne sono orgoglioso perché a quel tempo ne ero il produttore e, insieme ad Andrea Barbato, l'autore del testo. È stata una dimostrazione di problemi e di violazioni che in quel momento erano in corso perché è molto difficile tenere a bada un regista come Antonioni, quando gli si dà il permesso di filmare un Paese come la Cina, cioè con talmente tante facce, tanti aspetti e tanti percorsi che alcuni è riuscito a rappresentarne. Ed è stato quindi un fatto di estrema rilevanza dal punto di vista della denuncia delle violazioni dei diritti umani. Ecco perché accostarsi anziché scostarsi ha il suo vantaggio.

e con un *opposite* *number*: cioè, il filosofo Eco con un filosofo, lo storico Le Goff con uno storico e io con un giornalista o un comunicatore o un esperto di televisione. Potete immaginare che cosa ne è nato: una serie di incontri di questo genere hanno prodotto scintille, problemi, tensioni, aule svuotate, aule riempite, persone che ci sostenevano e persone che creavano un grosso antagonismo.

visitata da uno storico come Jacques Le Goff, di fronte a platee di cinesi, per quanto condizionate da quella situazione. Tutto questo per dire che più ci avviciniamo ‑ confermo e sostengo ciò che ho sentito dire dai colleghi, anche dell'opposizione, che il problema dei diritti umani è certamente al centro di tutto questo discorso - con l'intento di fare in modo che ci sia un intrecciarsi di rapporti, più possiamo contribuire a far sì che alcune cose accadano di meno e altre cose forse non accadano più. Possiamo essere agenti del nostro tempo. Credo che questo sia lo spirito dell'accordo che abbiamo appena ratificato,

personaggi liberi, quali sono gli scienziati del nostro Paese, si incontrano sì sui campi specifici di pertinenza degli *opposite* *numbers*, dei loro antagonisti, ma su materie che, essendo della scienza, sono della vita e che, essendo della vita,

si recheranno sul posto ad affermare per «n» volte nel corso di un anno l'impegno ad allargare lo spazio dei diritti umani, fino a riconoscerli a quel livello di civiltà a cui noi di tanto in tanto noi stessi ci illudiamo di essere giunti (e poi sappiamo o scopriamo che anche noi siamo in cammino e siamo tutt'altro che arrivati).

famosa questione dei terribili mercenari arabi del Darfur che fanno strage di donne e bambini). Quindi, cerchiamo di non appiattire la questione, che purtroppo è multidimensionale molto più che tridimensionale. In ogni circostanza In ogni circostanza in cui abbiamo la possibilità di attuare quella che, con grande intelligenza, Giovanni Paolo II aveva chiamato l'interferenza umanitaria, ogni volta che si schiudono percorsi

che non è di cooperazione, che so, militare, ma è di collaborazione scientifica e dunque tocca il cuore di quei rapporti che vorremmo poter approfondire per poi cambiare. *(Applausi

la materia, sia pure in modo indiretto, è stata già trattata per il precedente disegno di legge. Io condivido con animo sincero le preoccupazioni che sono state espresse prima ed ora circa il tema drammatico dei diritti umani in Cina. Chi vi parla non ha simpatie o condivide il regime interno della grande Repubblica popolare cinese. Qui si tratta di vedere se il nostro Paese prima di tutto ha un interesse oggettivo,

è tra i più avanzati e che oggi è, come tutti sappiamo e vediamo, sulla scena internazionale. In secondo luogo, è appunto attraverso l'intensificarsi

Risale ad un periodo in cui non c'era un Governo di sinistra o di centro-sinistra: c'era il Governo presieduto dal senatore Andreotti, il IV Governo Andreotti. Era il 1978 e ci fu allora - lo riconosco - una lungimiranza di quel Governo in certi aspetti della politica internazionale che oggi io credo dobbiamo cercare di far rivivere, sia pure nelle nuove condizioni, e se possibile ulteriormente sviluppare. Per questi motivi, insisto per l'approvazione di questo Accordo. Il Governo, naturalmente, ritiene che la ratifica di questa intesa sia importante. È importante per il nostro sistema economico, per il nostro sistema di impresa, che oggi vede, soprattutto nei settori ad alto contenuto tecnologico, la necessità di affiancare alle attività e agli investimenti economici una costante

nelle condizioni il nostro sistema universitario, i nostri istituti di ricerca e anche il mondo privato di poter migliorare e rendere più efficace ed efficiente la cooperazione scientifica e tecnologica fra Italia e Repubblica popolare cinese. I settori citati sono settori cruciali per lo sviluppo, per le biotecnologie, per le tecnologie dell'informazione, per la scienza di base, per le tematiche dell'energia e dell'ambiente. Sono settori cruciali e strategici e il

il nostro Governo ha posto costantemente il tema dei diritti umani. Abbiamo sempre tentato di affiancare alle grandi iniziative di promozione del nostro sistema economico e commerciale e alle opportunità che oggi è possibile cogliere in quel Paese puntuali richieste.

e il tempo di lunghe trattative sindacali; singoli imprenditori faranno sicuramente buoni a affari, e d'altra parte devono fronteggiare la concorrenza internazionale non soltanto propriamente cinese, ma anche degli altri Paesi che, a loro volta, investono e producono in

sento il bisogno di esprimere qualcosa di diverso; allora, va bene anche l'umorismo che è stato suggerito,

eseguire 500 condanne a morte l'anno, una decina la settimana; non credo che questo sia nulla e pertanto non ritengo che il ragionamento numerico valga. L'altro argomento che si attribuisce un po' scherzosamente - con un umorismo evidentemente amaro

i rapporti tra l'India e l'Italia sono intensi sia per quanto riguarda la ricerca, sia per quanto riguarda i rapporti tra le imprese, non soltanto perché in questo momento, tra l'altro, c'è una intensa attività del Governo, ma anche perché ci sono delle visite programmate anche da parte di Presidenti di Regione (cito la regione Campania e la regione Lombardia, con il presidente Formigoni). Del resto, l'India è un grande Paese per quanto riguarda la conoscenza: ci sono 380 università scientifiche e ci sono ogni anno 525.000 ingegneri laureati, è questo che fa dire che la prossima superpotenza della conoscenza sarà l'India. Ritornando al provvedimento cui lei ha fatto riferimento, mi rifarò alla relazione scritta. Desidero soltanto evidenziare tuttavia alcuni aspetti, perché è stato oggetto di particolare e intenso dibattito in Commissione Commissione Il provvedimento, prima di tutto, si rende necessario per dare attuazione legislativa ad un accordo che costituisce un preciso impegno politico assunto dal Governo italiano in materia di cooperazione con l'India nel settore della difesa, in un quadro di salvaguardia dei reciproci interessi in termini di miglioramento delle capacità militari nel campo dell'addestramento e nei settori tecnologico ed industriale. infatti riferimento, in modo particolare, al seguito degli impegni contenuti nel Memorandum d'intesa sulla cooperazione nel campo dei materiali della difesa, che è stato stipulato tra i due Paesi il 4 novembre 1994 e ratificato dall'Italia il 23 marzo 1998, con la legge n. 203. Dicevo, appunto, che questi sono gli elementi che costituiscono la cornice del provvedimento

e sono individuati in questo stesso articolo, in particolare, le categorie di materiali di armamento oggetto dell'eventuale scambio e le possibili modalità dello stesso.

impegna il Governo ad assicurare che nel rilascio delle autorizzazioni relative alle operazioni di trasferimento di armamenti sia previsto il concerto del Ministero degli affari esteri, in conformità

perché deve essere ovviamente applicata; soprattutto, voglio citarne l'articolo 1, che esprime il divieto al transito e all'esportazione di materiale verso i Paesi in stato di conflitto armato, che quindi sono in contrasto con i principi dell'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, verso i Paesi in cui la politica contrasti con i principi dell'articolo 11 della nostra Costituzione, verso i Paesi nei cui confronti sia stato dichiarato l'embargo e verso i Paesi in cui i Governi si sono resi responsabili di grandi violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti umani. Da ultimo, verso i Paesi che, in ragione dell'applicazione della legge n. 49 del 1987 sulla cooperazione, destinino nel proprio bilancio militare risorse eccedenti le esigenze di difesa del Paese. Ho voluto evidenziare questi aspetti perché il Parlamento vuole sottolineare in modo particolare che il Governo si attenga a queste misure; del resto, lo stesso Parlamento, da questo punto di vista, è nella condizione di poter poi verificare tutto quanto in ragione della valutazione che potrà fare, perché, come sappiamo, entro il 31 marzo di ogni anno il Governo è tenuto a presentare una relazione sulle operazioni effettuate nell'anno precedente.

Signor Presidente, mi pare quanto mai appropriato e opportuno un dibattito che coinvolga i nostri rapporti di *partnership* con l'India proprio in questi giorni in cui il nostro Paese, non il nostro Governo, è impegnato in uno sforzo in prima persona per rafforzare quei rapporti di *partnership* economici e commerciali con l'India e per diventare un punto di riferimento cruciale di quel tumultuoso e straordinario sviluppo economico che sta cambiando la faccia del contenente asiatico e di cui l'India è forse la prima protagonista. Di recente il presidente Prodi, presentando il suo viaggio in India su «Il Sole 24 ORE», ha fornito qualche dato dello straordinario sconvolgimento che è in corso in quell'area del mondo: l'India, che oggi rappresenta l'uno del PIL mondiale, lo triplicherà nel 2030 e raggiungerà nel 2050 la quota del 12 per cento del PIL mondiale, più dell'intera Unione Europea messa insieme. Nei prossimi cinque anni un quarto di tutti i nuovi posti di lavoro che verranno creati nel mondo verranno creati dall'India e, per gli appassionati di statistiche, si può concludere semplicemente dicendo che si calcola che nell'arco di 30 anni, cioè poco più di una generazione, l'India diventerà la terza potenza mondiale dell'universo. Ci troviamo di fronte a fenomeni e a dati che descrivono, con efficacia, un aspetto della globalizzazione che troppo spesso è sottaciuto o

cioè il valore straordinariamente progressivo di questo fenomeno di apertura dei mercati e anche di equità e di giustizia che sta sollevando dalla condizione di sottosviluppo e di miseria centinaia di milioni di persone sulla faccia della terra. Ciò dovrebbe consigliare ad un Paese come il nostro di non sopravvalutare gli egoismi economici e nazionali di fronte a fenomeni di portata così positiva e di non sottovalutare i vantaggi economici e commerciali che per un Paese ad avanzato sviluppo come il nostro e per l'Unione Europea nel suo complesso possono derivare. Per quanto riguarda l'India, va anche aggiunto che per fortuna qui non dobbiamo immergerci nel *grand guignol* che è stato in buona parte correttamente descritto a proposito della Cina perché parliamo della più grande democrazia del mondo. L'unico Paese

apprezzabili e benedetti dopo la drammatica e terribile tragedia del conflitto religioso che caratterizzò la partizione del 1948,

ad un Paese con queste caratteristiche e tradizioni, credo sia quanto mai opportuno un rapporto di *partnership* che riguardi anche la cooperazione militare. L'India può rappresentare un fattore di estrema ed enorme importanza nella stabilizzazione di un'area delicata e complessa nella vicenda mondiale, come l'Asia. Credo, infatti, come è ormai ampiamente dimostrato anche nelle vicende di questi anni, che l'opera di stabilizzazione e di pacificazione del mondo non possa avvenire senza l'impegno delle potenze regionali in ogni singola area regionale: il mondo si è rivelato troppo grande anche

in uno stato di guerra con il Pakistan per un conflitto relativo ai confini tra i due Paesi, ma, soprattutto, l'India è un Paese dotato di un arsenale atomico.

nel suo ruolo di promozione della democrazia dello Stato di diritto, dei diritti umani e della pace nel continente asiatico. A tal proposito, trovo perfettamente corrispondenti a queste preoccupazioni i due ordini del giorno che impegnano il Governo ad escludere dall'accordo le *cluster bomb* e le mine antiuomo, nonché, naturalmente, il riferimento, che in qualche modo

che abbiamo sviluppato nel dibattito precedente e pensiamo che oggi debba essere interrotta una continuità rispetto al passato che vedeva la cooperazione nel settore della difesa, in questo caso anche della vendita di armi, come una modalità prioritaria per la politica estera. Noi pensiamo che oggi sia necessario svolgere un'inversione di tendenza essendo profondamente convinti che l'Italia possa esportare tecnologie appropriate ad alto contenuto però certamente non utilizzando l'industria degli armamenti e il comparto industriale militare come volano per la ripresa economica e gli scambi commerciali. Per questo pensiamo che oggi con il nostro voto di astensione - dunque non un voto contrario

ci preoccupa la firma del *Memorandum* d'intesa sul *joint strike fighter*. Riteniamo che i posti di lavoro possano essere costruiti e moltiplicati attraverso la riconversione dell'industria bellica e che anche i rapporti tra Paesi grande rilievo per la democrazia come l'India, che può rappresentare anche il nocciolo fondamentale di un assetto multipolare, possano essere improntati verso un altro tipo di cooperazione, che veda nello sviluppo nello sviluppo sostenibile o comunque nella tecnologia eco-compatibile una delle chiavi di volta. L'India è oggi tra i principali produttori al mondo di carbone e di gas serra.

(IPCC), forse è possibile intervenire su quello, non continuando a pensare ad un modello di pacificazione continentale basato invece sulla forza delle armi. Approviamo e guardiamo con molto favore anche all'impegno preso dalla Commissione rispetto

una delle motivazioni addotte in Commissione esteri riguardava proprio il ruolo propulsore che l'Italia può svolgere in termini di rilancio dell'iniziativa diplomatica anche a livello regionale. Poco si comprende perché proprio oggi si debba ratificare un accordo militare con uno dei che invece deve essere un attore fondamentale per quel processo di pacificazione e di rilancio dell'iniziativa diplomatica per quanto riguarda un altro grande, grave e serio conflitto in Afghanistan.

sulla necessità di lavorare ad una riconversione dell'apparato produttivo del nostro Paese e certamente non ad un aumento delle spese militari e delle esportazioni dell'industria della difesa.

degli armamenti, che il problema del disarmo è da affrontare in maniera più seria e che dovremmo costruire una politica su questo tema. Tuttavia, in Commissione - ne abbiamo discusso attentamente e lo ricordava poco fa il senatore Pianetta

che intorno a questo scacchiere fondamentale ci debba essere un confronto sempre più aperto ed auspico che tale confronti passi dalle armi ad altri elementi importanti della scienza, della cultura e dello sviluppo

Signor Presidente, quando parliamo di politica estera e di politica della difesa accade spesso che quest'Aula scompagini un po' un po' le fila, nel senso che non si sa mai da che parte arriva il sostegno al Governo. Anche in questa occasione mi sembra non faccia specie che una parte della sinistra, quando soltanto sente l'espressione «militare», aprioristicamente deve dire di no e chiudere la porta.

con la Repubblica indiana. Non possiamo che essere estremamente favorevoli a tale accordo; da una piccola analisi, abbiamo potuto verificare

Valley, ma un distretto indiano, il distretto di Bangalore, dove tutte le multinazionali che operano nel campo dell'informatica hanno concentrato le loro produzioni e i loro studi. Stiamo parlando, in questa tornata, di rapporti italo-cinesi e italo-indiani. Sono i rapporti che caratterizzeranno probabilmente il nostro futuro e il futuro dell'umanità perché, sullo scenario internazionale, sono proprio queste due grandi potenze che si stanno affacciando con un'impressionante dinamicità. La grossa differenza tra i due sistemi è che quello cinese si basa su una bassissima tecnologia, sul manifatturiero, sostanzialmente sulla produzione di beni; viceversa, l'India si sta specializzando nella produzione di servizi e per di più servizi ad altro valore aggiunto, servizi che trovano radicamento nella scienza delle telecomunicazioni, nella scienza della tecnologia informatica. La prima spesa della famiglia media indiana è l'investimento nella scolarizzazione dei figli,

di alto valore non può che trovarci estremamente d'accordo. Ai colleghi che, viceversa, hanno votato con una certa disinvoltura le precedenti due leggi che ratificavano accordi con la Cina ricordiamo che il